La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 10 gennaio. L’ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 16, prevede la discussione del decreto-legge sulla governance del “Piano Mattei”. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19 di oggi. Mercoledì 20 dicembre, alle ore 12, sarà discusso il disegno di legge in materia di disposizioni sul made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19 di domani. Sempre mercoledì, alle ore 17, avrà inizio, anche ove non concluso il disegno di legge sul made in Italy, la discussione del disegno di legge di bilancio, che si articolerà secondo quanto stabilito dall’articolo 129 del Regolamento. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di domani. Nella giornata di giovedì 21 dicembre proseguirà la discussione generale del disegno di legge di bilancio e si procederà alla votazione degli articoli della seconda sezione del disegno di legge e degli eventuali emendamenti. Si passerà quindi all’esame della prima sezione del disegno di legge di bilancio. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo della prima sezione, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all’organizzazione del relativo dibattito. Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia che si svolgeranno venerdì 22 dicembre, alle ore 9,30, con trasmissione diretta televisiva. Una volta votata la fiducia, si riunirà la 5ª Commissione permanente per l’esame della Nota di variazioni. Seguirà quindi la votazione della Nota di variazioni e il voto finale del disegno di legge di bilancio, con la presenza del numero legale. Il calendario della prossima settimana prevede, se necessario, sedute a partire da martedì 27 dicembre, alle ore 17, e fino al 29 dicembre, per discutere l’eventuale seguito del disegno di legge sul made in Italy. Dopo le festività di fine anno, l’Assemblea tornerà a riunirsi martedì 9 gennaio, alle ore 17, con comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori. A tal fine, la Conferenza dei Capigruppo è convocata lo stesso giorno alle ore 16. È stato intanto stabilito che mercoledì 10 gennaio, previa convocazione della Giunta per il Regolamento, sarà discusso il documento di riforma del Regolamento del Senato recante l’introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura. Per la votazione in Assemblea è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. È stato inoltre previsto l’inserimento, nel calendario della settimana del 16 gennaio, del disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario nonché del disegno di legge costituzionale, di iniziativa popolare, di modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione. La Conferenza dei Capigruppo ha altresì convenuto di confermare nella sessione annuale del 2024 la delegazione dei senatori attualmente in carica presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.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

n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano (936) La seduta è tolta